ribadisco quanto, a nome del mio Gruppo, ho espresso in Conferenza dei Capigruppo. Siamo in Aula oggi per una *fictio*, per la rappresentazione di una realtà che non sarà quella che si svilupperà nei prossimi minuti, nelle prossime ore e nella giornata di domani. Ci troviamo, nonostante le smentite di autorevoli esponenti di Governo e di autorevolissimi esponenti della maggioranza, anche del Senato, di fronte all'ennesima richiesta di fiducia su un provvedimento che noi avremmo voluto e dovuto discutere insieme per migliorarlo. Quando il ministro Tremonti, una settimana fa, venne in Commissione e ci rifilò un articoletto in cui parlava di manette agli evasori, gli dicemmo era un testo insufficiente, e pensavamo che sarebbe arrivato qualcos'altro. Ci fu risposto che quello era il testo definitivo del Governo, su cui il Parlamento sarebbe stato chiamato a discutere. Oggi, invece, come apprendiamo prima dalle agenzie e come è stato confermato poi dal Governo nella Conferenza dei Capigruppo - ormai la prassi parlamentare va cambiando, e le notizie e i lavori parlamentari vengono dettati

ho davvero paura che si stia scherzando con il fuoco. Il Paese, come dimostra la manifestazione di questa mattina, in grande difficoltà, con grande sbigottimento e con grande preoccupazione ma con estrema determinazione, chiede al Governo e al Parlamento di adottare misure eque e giuste, che siano in grado di rassicurare, innanzitutto gli italiani e immediatamente dopo i mercati. L'Italia dei Valori non accetta che si facciano degli aggiustamenti meramente contabili sulle spalle degli italiani. Per questo avevamo chiesto a lei, signor Presidente, di evitare di incardinare il provvedimento questa questa sera, perché incardiniamo un provvedimento che non sappiamo domani, dopo la presentazione del maxiemendamento del Governo, su quali basi si fonderà. É anche una mancanza di rispetto nei confronti

assolutamente fondati sulle palafitte ed essere quindi caducati dal maxiemendamento del Governo. Ringrazio anche lei, Presidente, perché fin dall'inizio ha

occorre fare in modo che la manovra venga approvata al più presto (e colgo l'occasione proprio di questa seduta per ringraziare pubblicamente tutti i componenti della Commissione bilancio del Senato, i quali con grande spirito di abnegazione e senso di responsabilità hanno instancabilmente lavorato, anche per tutta la giornata di domenica, per esitare il provvedimento che è oggi all'esame dell'Aula). Verosimilmente parte di questo provvedimento potrà essere modificata, ma questo fa parte della fisiologia parlamentare: le regole sono queste. Chi come me in passato aveva cercato di esorcizzare il voto di fiducia,

Presidente, mentre il Senato si interroga sulla presentazione o meno di un maxiemendamento da parte del Governo, tutte le forze responsabili dell'economia, delle istituzioni e della politica in Europa si chiedono che cosa stia facendo l'Italia. Oggi abbiamo assistito a delle prese di posizione da parte del maggior Paese dell'Unione europea, la Germania, che associano in modo molto preoccupante ed addirittura inquietante la situazione economico-finanziaria dell'Italia a quella della Grecia.

il portavoce del Governo spagnolo, di un Governo che a causa della crisi ha annunciato le proprie dimissioni e ha convocato nuove elezioni - la criticità e la delicatezza della situazione in cui si trovano i mercati e gli investitori per le incertezze italiane.

siamo grati anche per aver detto a più riprese che il suo obiettivo e quello di quest'Aula era e doveva essere di consentire un esame di merito e la possibilità di un miglioramento dello stesso da parte del Senato della Repubblica. Lei, signor Presidente, ha detto un istante fa che questa manovra va approvata al più presto; penso che i colleghi siano consapevoli che una cosa sono i tempi e una cosa è il merito di questa manovra.

dal Capo dello Stato, non era un richiamo alla tempistica nell'approvazione della manovra, ma alla qualità della manovra, alla credibilità della manovra, poiché arrivano ai vertici delle nostre istituzioni, signor messaggi inequivocabili sulla preoccupazione relativa al fatto che l'Italia stia ballando su un baratro senza adottare misure adeguate. Ogni giorno e ogni ora, si può dire, le agenzie battono notizie su come questa manovra debba essere rifatta. Segnalo a colleghi relativamente distratti che la notizia diffusa dal Governo, secondo cui si annuncerebbe una imposizione del 3 per cento su redditi o patrimoni superiori a 500.000 euro,

dell'annuncio di misure straordinarie, come patrimoniali e misure sull'evasione fiscale, che arrivano e spariscono. Infine, signor Presidente, noi non sappiamo ancora se stasera, come lei ha ricordato correttamente, il Governo presenterà il suo maxiemendamento oppure no e, dunque, se noi ci troveremo, domani mattina, a riaprire l'Aula del Senato senza neppure sapere se la quarta o quinta manovra, da luglio e poi da agosto, sia stata effettivamente approvata dal Consiglio dei ministri. In passato, signor Presidente, ricorreva la celebre espressione, tante volte richiamata in quest'Aula, che "mentre a Roma

non credo che voi possiate fare gli spiritosi, perché dovete dirci se siete disponibili a misure sulla previdenza, se siete disponibili a tagli della spesa pubblica, se siete disponibili a misure reali, e non figurative, per il contrasto dell'evasione fiscale. Questo chiedono i mercati, le istituzioni finanziarie e l'Europa! Qui ci si continua a consultare. Il Senato non potrà discutere, ma dovrà affrontare una

i suoi effetti sarebbero stati rimangiati; la manovra di agosto è già stata divorata dai mercati. Da qui a domani mattina, se la maggioranza e il Governo non si pongono nelle condizioni di dire la verità agli italiani,

dovrebbero invece dare un messaggio al Governo di risolutezza e di coraggio. Qui c'è un'opposizione che ha dichiarato di essere pronta, stando all'opposizione, a votare misure, anche difficili ed impopolari, ove fossero strutturali e credibili. Abbiamo la sensazione che stiamo andando verso la quinta manovra, destinata a vedere poi l'arrivo della sesta, della settima, e che ci inoltriamo in un precipizio senza fine. Mi auguro che non sia così, signor Presidente, ma stiamo discutendo di questo. E mi auguro, infine, che non si inizi l'esame di una manovra che non c'è più, la si incardini formalmente, che il relatore dica una parola che rimandi alla presentazione del maxiemendamento: abbiamo la dignità di non fingere di svolgere in questa sede un dibattito su una manovra che già non c'è più, perché non sarebbe dignitoso se il Parlamento fingesse di esaminarla!

In quella occasione il presidente Berlusconi in quest'Aula ebbe modo di illustrarci il fatto che il sistema era sano, le banche solide, le famiglie floride, le imprese in pieno sviluppo, la disoccupazione calante. I giorni successivi registrarono un perturbamento gravissimo dei mercati finanziari, un turbamento che si estendeva ai titoli di Stato italiani in maniera assai sensibile, la preoccupazione vivissima della BCE e degli altri Paesi europei e l'inizio di quella faticosa e dolorosa attività attività di acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca centrale europea che valesse a salvaguardare - nella misura in cui poteva farlo dalla tempesta il nostro debito pubblico. Quell'attività, peraltro, è continuata a tal punto che oggi è ingentissimo l'impegno finanziario che la BCE ha investito sui titoli italiani.

sta ponendo l'Italia in una situazione oggettivamente critica, tanto che la riunione del direttivo della BCE di giovedì viene attesa con particolare preoccupazione per la ragione che in esso maturerà anche la decisione se continuare o meno ad acquistare i titoli di Stato italiani. Dico

probabilmente tutto ciò che sta accadendo in queste ore ci sembrerebbe del tutto inspiegabile, una favola amara, una sorta di *fiction* per tenere occupato il Senato. Ma c'è di più. Spinto dalla erroneità tragica delle parole pronunciate al Senato e alla Camera, l'11 agosto, cioè esattamente otto giorni dopo, il Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi vara una manovra finanziaria, che approda immediatamente al Senato e che è stata oggetto dell'esame da parte della Commissione bilancio. Ma c'è di più. Questa manovra finanziaria ha mutato continuamente anima e pelle nel corso di queste settimana nelle quali la Commissione bilancio ha ininterrottamente lavorato su testi continuamente diversi. Ne sono rimaste identiche tre caratteristiche: il fatto di non contenere misure strutturali, il fatto di non avere misure per la crescita, il fatto di essere fortemente iniqua nelle misure che sono state scelte. Ma soprattutto soprattutto rimane il giudizio che abbiamo ininterrottamente ripetuto in queste settimane: questa manovra non è sufficiente; questa manovra non rende credibile l'Italia, questa manovra non aiuterà il Paese a uscire dal guado, non cambierà il giudizio dei mercati e degli osservatori Ma lo sforzo dell'opposizione, di cui ormai tutti ci danno atto, sta non soltanto nel fatto di aver detto la verità sin dal primo momento - come sin dal primo momento dicemmo la verità sulla crisi - ma anche nel fatto che che abbiamo continuato a lavorare attendendo pazientemente, da idea balzana a idee balzane, da *summit* a consigli vari, a luoghi di riunione, ad eremi di Lorenzago, a rientri in campo del Ministro dell'economia, dall'abolizione delle pensioni di reversibilità alle limitazioni del del conteggio ai fini pensionistici degli anni di università. Ne abbiano sentite di tutti i colori, e nel frattempo il tempo trascorreva. Quindi quell'urgenza, talmente drammatica e pressante da far cambiare così radicalmente l'opinione e l'agire del Presidente del Consiglio dal 3 agosto all'11 agosto, ci porta ad oggi perché il Governo e la sua maggioranza non sono stati in grado di appianare fra di loro le controversie e di presentare una manovra avente le caratteristiche che ci richiede il momento e i soggetti di cui ho parlato. Nel frattempo l'opposizione contribuiva con le sue proposte. Era in grado di essere puntualmente disponibile ad ogni nuovo incontro, ad affrontare ogni nuovo tema e ad approvare la manovra entro domani. Ora vorrei che fosse chiaro che questo ci costa davvero molto, anche perché tra i grandi assenti di questi giorni c'è la politica. Lo dico con un accenno e ne parleremo poi domani. Ma vi pare normale che in un Paese che si trova in questa gravissima situazione un Governo, che è così indeciso e - lasciatemi dire - pasticcione e rissoso, e che trova dall'altra parte opposizioni serie, responsabili, propositive e puntuali, ha come unico mantra giornaliero infilare due dita nell'occhio alle opposizioni? Mi chiedo quale sia il senso politico di questa cosa. Così come mi chiedo perché in una situazione come quella attuale, visto che non porta una lira nelle casse dello Stato, bisogna mantenere una norma, l'articolo 8, che spacca il Paese e porta milioni di persone in È inspiegabile, se non iscritta nell'assoluta inadeguatezza del Governo ad affrontare questa fase.

diventa il *totem* entro il quale far entrare il voto di fiducia su misure che colpiranno comunque il Paese. Ora non discuto dell'esattezza delle manovre perché non le conosco, perché nessuno si è peritato di informare le opposizioni responsabili di che cosa bolle in pentola, perché immagino che il livello di confusione e di tensione dentro al Governo e alla maggioranza sia molto alto.

sia particolarmente grave. Presidente, lo dico con l'attenzione e la responsabilità con la quale fino a questo momento ci siamo comportati. Com'è che il Governo non riesce a comprendere che una manovra adottata nella pienezza dell'esame da parte del Parlamento, comunque vada il voto, dà il senso di un Paese che vede pienamente coinvolte le istituzioni rappresentative nell'esame e nell'adozione di una manovra? È un'ulteriore debolezza. Non comprendere queste *nuance* - me lo lasci dire e aggiungo che *nuance* non sono, bensì elementi strutturali di definizione della questione politica mi pare significhi - questa è l'impressione che avranno anche i cittadini italiani - che il Governo sin dall'inizio è assai più attento a salvarsi dalle tensioni interne che a pensare al bene dell'Italia. *(Applausi dai

sera. Comprenderà però, signor Presidente, che, per quanti sforzi si facciano, la preannunziata questione di fiducia a tutti è imputabile tranne che ai Gruppi d'opposizione; ricorderà infatti che già una settimana fa, quando in Commissione bilancio sono stati depositati circa 1.300 emendamenti, di cui 700 della maggioranza, noi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a ritirare

mesi e che c'è un contesto nazionale ed internazionale particolarmente complesso, comprenderà che, almeno in questa fase, che si presenta estremamente delicata, dobbiamo comunque

in gran parte diverso da quello esaminato e votato dalla Commissione bilancio, compresi gli emendamenti, sostanzialmente modificativi del testo originario, che il Governo ha presentato «a rate» nel corso della discussione in Commissione. Ora, se così è, comprenderà che valutare misure come l'aumento dell'IVA (che non si comprende come si concilierà con la questione della riforma fiscale, perché si diceva che non si poteva aumentare perché doveva essere una sorta di

è così o meno e quale sarà la platea dei contribuenti che saranno interessati da questa discussione,

io eviterei di affrontare un dibattito ed una discussione generale su un testo, quello della Commissione bilancio, che è stato già preannunziato sarà cambiato dal maxiemendamento, perché delle due l'una: o il maxiemendamento conterrà delle novità sostanziali, così come ci è parso di capire anche dalla discussione che c'è stata ai più alti livelli delle nostre istituzioni, e quindi credo sarebbe corretto che i colleghi senatori senatori possano essere messi nelle condizioni di discutere di ciò che realmente sarà la manovra, o, viceversa, il maxiemendamento non conterrà quelle modifiche o quelle novità così importanti. Questa cosa da un certo punto di vista ci preoccupa ancora di più, perché significherebbe allungare una sorta di agonia, a cui, purtroppo, la maggioranza in queste due settimane ci ha aiutati e costretti. Signor Presidente, e concludo, un'amara considerazione noi la facciamo e credo che questa sia la cosa più grave e anche, dal nostro punto di vista, più seria per le valutazioni di carattere politico.

dalla lotta all'evasione fiscale. Il Ministro dell'economia ha così certificato che si trattava di una manovra ancora più forte, ancora più robusta, ancora più coperta e ancora più credibile di quella precedente. Prendiamo atto oggi Prendiamo atto oggi che il Governo ritiene non sia così, che questa manovra non sia coperta e non abbia quella autorevolezza che ci è imposta dagli obblighi comunitari.

questo Governo e questo Ministro dell'economia non abbiano le idee chiare su come si tengono in ordine i conti dello Stato. Se si cambia la copertura ogni settimana e poi si scopre che quella copertura non va bene, non è credibile e non garantisce la solidità della presenza economica del nostro Paese in Europa, credo che primi a trarne le conclusioni dovrebbero essere i colleghi della maggioranza e il Governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio.

questa manovra in pochi giorni in pieno agosto e si è subito dichiarato disponibile ad intervenire per migliorarla nella discussione parlamentare.

presentati anche dall'opposizione. Quindi è stato fatto un grande lavoro per migliorare il testo approvato dal Consiglio dei ministri. (e lo dico al presidente D'Alia, che è appena intervenuto dicendo che il Governo non ritiene corretti i saldi e, quindi, non ritiene corrette le coperture), non solo il Presidente della Repubblica, ma anche gli altri Paesi europei chiedono di inserire nuove norme strutturali al fine del contenimento del debito pubblico. Il che è proprio quello che stiamo per fare. Prima il senatore Rutelli diceva che i mercati ci stanno guardando. È vero, lo dico anche alla senatrice Finocchiaro: i mercati ci stanno guardando e hanno visto bene dove eravate voi oggi. Voi oggi, invece di essere in Parlamento a discutere della manovra, eravate in piazza con la CGIL...

Non solo eravate in piazza con la CGIL, ma mentre i mercati ci chiedono un'approvazione veloce di questo provvedimento, il segretario di un partito autorevole dell'opposizione, l'Italia dei Valori, l'onorevole Di Pietro, oggi ha parlato di ostruzionismo duro per bloccare la manovra al Senato. tutte le opposizioni hanno presentato più di 400 emendamenti alla manovra: alla faccia della volontà di concluderla in tempi brevi! Dunque, bene ha fatto il Governo

La simpatia personale che nutro per il presidente Bricolo mi consente di dirgli che questo intervento, secondo me, non serve al momento e ad un sistema di relazioni parlamentari corrette.

il Terzo Polo aveva prodotto iniziative ragionevoli, che confermiamo questa sera (c'è una nota ufficiale che richiama la maggioranza alla responsabilità verso il Paese), che riguardano: il sistema pensionistico; un'imposta patrimoniale seria, strutturata, misurata nei numeri, ma continua per garantire un flusso certo, da incrociarsi con la la vostra tanto dichiarata lotta all'evasione, che può diventare uno strumento per acquisire elementi aggiuntivi al gettito dell'erario; scelte precise in materia di liberalizzazioni e privatizzazioni. vi erano i contenuti di un incontro possibile, ragionevole, nell'interesse del Paese tra una maggioranza e un'opposizione responsabili. Ma non siete in queste condizioni. E sapete qual è Che ne siete consapevoli, perché individualmente sapete di una debolezza politica che parte dalla *leadership* politica della vostra coalizione, e dovete subire anche questa condizione parlamentare avvilente, perché non avete la forza di porre politicamente la questione della vostra responsabilità verso il Paese. *(Applausi dai Gruppi* Signor Presidente, credo che a nessuno sfugga la delicatezza e l'importanza dei momenti che stanno vivendo non solo l'Italia ma tutta la comunità internazionale sul fronte economico. Non voglio fare un intervento nel merito, che si farà in altra nelle prossime ore, ma credo che non possa nemmeno eludere i temi che alcuni colleghi hanno posto. Voglio, in primo luogo, dare atto al Governo di avere agito con tempestività. Non voglio aprire polemiche, lo cito come un fatto storico: tutti possono aver sbagliato valutazione, il Governo ma anche le opposizioni. Ricordo le dichiarazioni dell'onorevole Bersani che, quando si varò il decreto di luglio, propose - come riportato sui giornali e sulle agenzie

ai livelli europei la sollecitazione agli Stati membri di garantire l'azzeramento del *deficit* nel 2014 è stata anticipata, come richiesta, al 2013 (questi sono fatti storici che saranno sicuramente ricordati negli annali, perché non stiamo vivendo momenti ordinari), il Governo Berlusconi ha varato con grande rapidità e sollecitudine, in un contesto di confronti, sinergie e anche discussioni - perché no? - internazionali, un ulteriore provvedimento,

il Senato ha avuto l'onore e l'onere di lavorare; lo abbiamo fatto tutti (maggioranza e minoranze) durante il mese di agosto, senza alcuna esitazione o pausa, anche per dimostrare al Paese la serietà delle istituzioni, alle quali la si dovrebbe riconoscere. Dal 22 agosto le Commissioni hanno dato i loro pareri, la Presidenza la Presidenza del Senato ha garantito a tutti possibilità di espressione e abbiamo fatto una discussione nella Commissione bilancio. Io non faccio parte della 5ª Commissione, ma come Capogruppo ho seguito il lavoro dei colleghi, e li ringrazio tutti già ora, siano essi di maggioranza o di minoranza, per il lavoro svolto. Sono state approvate numerose modifiche: credo che in Aula siano arrivati oltre 60 emendamenti, di maggioranza e minoranza, che la Commissione ha approvato. Il presidente Azzollini e tutti i colleghi hanno svolto un grande lavoro. C'è stata capacità di ascolto. Voglio ringraziare il Presidente del Senato per le sue continue sollecitazioni a un confronto aperto tra maggioranza e minoranza e dargli atto di aver assunto, come sempre e più di sempre, vista l'emergenza del momento, una funzione *super partes* partes* e di garanzia anche rispetto alla questione della fiducia. Sinceramente gli auspici del Presidente del Senato sono stati pubblici, ripetuti e certamente sinceri, e tutti abbiamo condiviso l'auspicio di un confronto che non avesse la necessità della fiducia. Quando nelle ultime ore gli esponenti dei Gruppi di minoranza hanno pubblicamente dichiarato di essere disponibili a votare il provvedimento entro la giornata di domani, anche in funzione dei calendari internazionali che scandiscono le nostre decisioni (sono oggi centrali lo *spread* tra i titoli pubblici italiani e i *Bund* tedeschi e le decisioni della Banca centrale europea, europea, che giovedì avrà una riunione, ed è forse questa la scadenza che scandisce in questo momento i tempi dei Parlamenti), il presidente Schifani ha auspicato un dibattito senza fiducia, un confronto libero e franco, come in Commissione c'è stato. Anche sulle cifre - questo lo diranno i colleghi nel merito - la manovra è stata rinforzata durante l'esame in Commissione bilancio sia per le proposte venute dalla maggioranza e dal Governo che per le proposte venute dalle minoranze. Ho qui un foglio distribuito in occasione di una conferenza stampa del Partito Democratico dove ci sono alcune

Correttamente il Ministero dell'economia nel dare il parere positivo ha quantificato in zero questo rafforzamento della manovra perché è una eventualità e non possiamo oggi dare per certe delle cifre, ma io mi auguro che le valutazioni dei proponenti sui 10 miliardi di minore spesa siano reali perché vorrebbe dire avere una manovra ancora più salda.

Mi auguro sinceramente che questi due emendamenti tra i tanti approvati garantiscano 10 miliardi di minori spese e 4 miliardi di maggiori entrate: vorrebbe dire rinforzare i saldi della manovra di 14 miliardi di euro. Ma credo che le valutazioni prudenziali del Governo siano logiche, proprio per essere maggiormente

Potrei fare molte citazioni delle critiche di importanti *leader* delle minoranze al contributo di solidarietà o ad altre misure che poi sono state omesse. Le ho lette e sentite dai diretti interessati o nelle televisioni. Se la maggioranza si chiude a riccio è arrogante; se si apre alle modifiche se ne dia atto.

la Banca centrale europea (tutti guardiamo a questa scadenza, all'acquisto dei titoli e a tutto ciò che avviene sui mercati), c'è stato il richiamo autorevolissimo che nelle ultime ore è venuto dal Presidente della Repubblica che ha invitato a rafforzare la manovra e ovviamente - credo sia scontato - a rispettare i tempi, oltre che i saldi;

introduca misure di rafforzamento e scelga la via della fiducia, che noi tutti avremmo voluto evitare. Il nostro Gruppo, infatti, aveva presentato uno o due emendamenti, che era pronto a ritirare. Quindi, c'erano tutte le condizioni per una discussione senza il voto di fiducia. Credo che gli autorevolissimi richiami giunti, la necessità di garantire i tempi e le ulteriori misure di rafforzamento della manovra che saranno introdotte portino a questa decisione, di cui prendiamo atto, ringraziando - ancora una volta - il presidente Schifani e tutti coloro che hanno operato perché il dibattito si svolgesse - come di fatto si è svolto - in Commissione senza condizionamenti e nella capacità e possibilità di modificare la manovra. Non voglio fare polemiche: c'è il diritto di sciopero, ma c'è anche il diritto della maggioranza di definire sbagliati e intempestivi alcuni scioperi che - difatti - hanno trovato scarsa adesione nella

che, dall'una all'altra sponda dell'oceano, sta travolgendo l'Occidente. Nei giorni scorsi il presidente Obama ha dovuto accantonare i programmi ambientalisti che erano stati uno dei motivi vincenti della sua campagna elettorale (immagino lo abbia fatto con dolore), perché le aziende non potevano sopportare

dove sono stati licenziati 16.000 appartenenti alle forze dell'ordine: misure che l'Italia nemmeno osa immaginare, perché abbiamo bisogno di sicurezza. È un momento difficile, e la maggioranza lo affronterà con il senso del dovere che da sempre la caratterizza. Mi auguro che da tutti i settori del Parlamento non ci siano insulti, e non voglio enfatizzare

Al termine della discussione generale, ove non dovesse essere pervenuto l'emendamento del Governo annunciato in Conferenza dei Capigruppo, così come già deciso in tale sede, la seduta verrà tolta, per essere aggiornata a domattina alle ore

Onorevoli colleghi, le ultime settimane sono state - e sono tuttora - contraddistinte da una continua e, per qualche verso, irrazionale fibrillazione dei mercati finanziari in tutti i Paesi sviluppati, originata da movimenti finanziari che hanno interessato tutti i titoli in listino dei Paesi ritenuti - non sempre a ragione - come quelli...

Colleghi, per cortesia, movimenti finanziari che hanno interessato tutti i titoli in listino dei Paesi ritenuti - non sempre a ragione - come quelli maggiormente esposti a rischi di *default* della finanza pubblica. La forte volatilità delle quotazioni che ha caratterizzato il trascorso mese di agosto sembra anche segnalare il possibile inizio di una nuova fase di rallentamento per l'economia globale. Di conseguenza, appare sempre più urgente il rafforzamento dei meccanismi della *governance* globale degli stessi mercati finanziari affinché le fluttuazioni non si riflettano irrimediabilmente sull'andamento delle economie reali. gli elevati ed altamente volatili prezzi del petrolio e di altre materie prime, unitamente ad altri fattori, tra i quali rivestono particolare rilevanza la crisi dei debiti sovrani in Europa e l'incertezza sulla sostenibilità delle finanze pubbliche statunitensi, contribuiscono a creare un clima di sfiducia tra imprese e famiglie in tutto il mondo. Per ciò che riguarda l'area euro in particolare, la strategia usata da parte dei Governi europei nella gestione della crisi greca e la forte esposizione ai titoli di Stato greci da parte di molte banche francesi e tedesche hanno alimentato tensioni e sfiducia sui mercati finanziari, tanto da contagiare anche economie solide come la nostra. Qualora le economie avanzate subissero il brusco rallentamento atteso dai mercati finanziari, si accentuerebbero ulteriormente le differenze, in termini di potenziale di crescita, fra Paesi emergenti ed industrializzati, fenomeno che per certi versi appare comunque inevitabile nella prospettiva di lungo periodo. La forte integrazione delle economie nazionali e la stretta correlazione tra attività economica e solidità delle finanze pubbliche costituiscono pertanto la cornice epocale in cui inserire necessariamente i nostri problemi di competitività. Le tensioni sui mercati del debito italiano possono ridursi solo conferendo maggiore certezza al percorso di risanamento, ovvero se le prospettive di crescita dell'economia globale dovessero migliorare o qualora si riducessero i margini di incertezza relativa alla crisi dell'euro. L'evoluzione degli scenari economici ha pertanto indotto il Governo ad intervenire urgentemente con un'ulteriore manovra correttiva di rafforzamento ed anticipazione degli effetti del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio già nel 2013, anziché solo nel 2014, come era stato inizialmente previsto e concordato in sede comunitaria. È noto che il Governo ha deciso oggi di rafforzare ulteriormente questa manovra,

di ciò che potrà contenere l'annunciato maxiemendamento del Governo, la manovra che ci apprestiamo ad esaminare registra interventi pari a 47 miliardi di euro nel biennio 2012-2013, in conto minori spese e maggiori entrate, per lo più volte all'anticipazione del rafforzamento di misure già adottate con il decreto-legge n. 98 del 2011. I maggiori effetti di contenimento della manovra integrativa tendono a concentrarsi nel biennio 2012-2013 per anticipare il pareggio di bilancio in quest'ultimo anno. La manovra netta porta ad un miglioramento del saldo, in termini di indebitamento netto, di circa 18 miliardi nel 2012, 25 nel 2013 e di oltre 7 nel 2014 ed effetti simili si registrano in termini di fabbisogno. Marginale è invece l'effetto nel 2011, per il quale si registra un miglioramento dei tre saldi per circa 31 milioni. Il contenuto del provvedimento, nelle sue linee portanti, è ampiamente noto: si interviene sia sul lato della spesa, con misure di razionalizzazione, che sul lato delle entrate, essenzialmente con misure di ricomposizione del gettito in direzione delle agevolazioni oltre che con decise misure di contrasto all'evasione. Più nel dettaglio, al Titolo I, all'articolo 1, comma 1, si incrementa 1'accantonamento di risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato per gli anni 2012 e 2013. L'articolo stabilisce poi per le amministrazioni centrali anche una riduzione delle dotazioni organiche, dirigenziali e non, del 10 positivi ai fini dell'indebitamento netto previsti in termini di riduzione delle deduzioni ed agevolazioni fiscali dall'articolo 40, comma 1-*quater*, primo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono anch'essi anticipati agli anni 2012 e 2013, prevedendosi un effetto pari a

dall'articolo 20 della manovra di luglio, oltre ad anticipare, a decorrere dall'anno 2012, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con riferimento ai parametri di virtuosità previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011. Per quanto concerne il capitolo della previdenza, fermo restando sempre quanto eventualmente dovesse contenere

comma 21 armonizza le regole di decorrenza del pensionamento del settore della scuola, in precedenza escluso, a quello degli altri settori produttivi, tenendo conto della specificità programmatoria del settore. Le disposizioni indicate ai commi 22 e 23 sono poi dirette ad introdurre misure di posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per il pensionamento di vecchiaia o per limiti di servizio. In tema di entrate, sull'articolo 2 va segnalata la previsione che affida al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione di tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, con la possibilità di introdurre, tra l'altro, nuovi giochi, indire lotterie ed adottare nuove modalità di gioco del Lotto. Con il comma 4, si riduce ulteriormente il limite di utilizzo legale dei contanti come mezzo di pagamento, portandolo a 2.500 euro. Le norme previste ai commi a 34 sono poi finalizzate all'adozione di un'aliquota unica, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento, attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari. Il comma 35 interviene poi sulla limitazione della potestà accertativa nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore. Il comma 36 prevede infine che le maggiori entrate derivanti dal decreto siano riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria. Al Titolo II, in tema di misure per favorire lo sviluppo, si segnala l'articolo 3, che reca norme volte a ridurre gli oneri amministrativi e procedimentali, talvolta eccessivamente onerosi, che oggi limitano la libertà di impresa, impresa, e a favorire il rilancio dell'economia. Vanno inoltre segnalati: l'articolo 4, che introduce varie disposizioni volte alla piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica imponendo norme in grado di creare le migliori condizioni per l'apertura al mercato di tale settore strategico per la crescita economica; l'articolo 6, che reca misure in tema di semplificazione e razionalizzazione della segnalazione certificata di inizio attività, denuncia denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione; l'articolo 7, che apporta modifiche alla disciplina delle fonti rinnovabili. Rispetto al testo del decreto-legge, la Commissione ha approvato numerosi emendamenti, accogliendo l'invito del Presidente del Senato a non guardare la firma dei proponenti. Si tratta frutto di un lavoro intensissimo, che ha visto impegnati tutti i commissari in un'instancabile attività di approfondimento e di proposta. Ne sono sortite molte proposte certamente migliorative, sia sotto il profilo della tenuta dei saldi finanziari che della concreta attuabilità delle misure contenute nel decreto-legge Elemento imprescindibile del lavoro della Commissione è stata l'esigenza di mantenere invariati, e semmai di migliorarli, i saldi della manovra. Dai lavori della Commissione bilancio, tali saldi escono decisamente rafforzati grazie ad una serie di norme introdotte nel corso del dibattito. meritano una menzione particolare quella sul recupero delle rate non pagate del condono del 2002, la normativa riguardante la *spending review* infine le misure attinenti ai *money transfer*. Sul fronte delle minori risorse, è stata invece decisa la soppressione del contributo di solidarietà e una significativa riduzione dei tagli per gli enti locali.

determinando così un miglioramento dei saldi, sia per competenza sia per cassa. Per quanto concerne il disegno di legge di conversione, è stata inserita una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari: l'intento è quello di realizzare risparmi di spesa e un incremento di efficienza, con l'osservanza di una serie di principi e criteri direttivi volti alla riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, delle sezioni distaccate e alla ridefinizione altresì dei distretti di corte d'appello. Le modifiche più rilevanti prevedono dunque l'alleggerimento dei tagli sugli enti e la soppressione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, i loro effetti sono ampiamente compensati dagli interventi di contrasto all'evasione, dall'implementazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari e dalle misure stringenti in tema di società di comodo. Per quanto riguarda gli enti locali, va sottolineata la previsione dell'attribuzione dell'intera quota delle risorse derivanti dagli accertamenti tributari da loro attivati. attivati. Circa la lotta all'evasione, è stato mosso un rilievo in ordine all'inopportunità di ascrivere rilevanti effetti di maggiore entrata alle norme repressive dei comportamenti fiscali illeciti.

Dunque, le misure che nel decreto-legge in discussione sono state identificate partitamente ben possono conseguire e forse migliorare i risultati che ci si prefigge. Per quanto concerne le maggiori risorse, esse deriveranno dagli emendamenti in tema di contrasto a fenomeni non solo evasivi ma anche elusivi. Mi riferisco, in particolare, alle norme in tema di società di comodo e di *trust*, come ho già alla riduzione della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi della quota degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria. Signor Presidente, va sottolineato che nel corso dei lavori non è mancato, anzi è stato prezioso, l'apporto - certo talvolta critico, ma sempre costruttivo - dell'opposizione, circostanza che ha determinato anche l'approvazione di importanti proposte

L'emendamento prevede, dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, interessati, presenti al Parlamento, entro il prossimo 30 novembre, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede, in particolare, in coerenza con quanto linee guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale,

L'impatto che un simile programma di riforme può avere per il prossimo futuro sull'organizzazione amministrativa è di tutta evidenza. Al Ministero dell'economia è pertanto affidato il compito di definire i costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. A ciò dovrà conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013. Ovviamente, il Parlamento rimane il *dominus* dell'intero processo, essendo richiesta l'espressione del parere da parte delle Commissioni sui decreti di variazione conseguenti alle rimodulazioni di spesa funzionali alla maggiore flessibilità di bilancio. Signor Presidente, colleghi, l'occasione dell'esame di questo provvedimento rende possibili alcune brevi considerazioni. Nel complesso va nuovamente assicurato che la manovra contenuta nel decreto in esame presenta un sicuro effetto di correzione dei saldi tendenziali, permettendo il raggiungimento del pareggio già nel 2013. Va sottolineato, al tempo stesso, che il vero tema centrale di politica economica di oggi, che fa da sfondo anche alla questione, critica già da anni, su come assicurare la sostenibilità della finanza pubblica nel medio periodo, è quello di elaborare tutte quelle misure che siano idonee a favorire l'accelerazione del tasso di crescita dell'economia. Esso infatti si pone oggi in Italia su livelli che sono ancora inferiori a quelli che in media si registrano negli altri Paesi sviluppati. L'urgenza del contesto rende però necessario riconoscere oggi distintamente, con lucidità in termini prospettici per i prossimi anni, gli effetti di retroazione che gli andamenti e le manovre sulla finanza pubblica generano di volta in volta sull'economia, e nondimeno, soprattutto, distinguere con chiarezza i riflessi che gli andamenti di quest'ultima inevitabilmente producono anche sulla prima. Ebbene, tale profilo costituisce oggi, oltre che un tema antico del pensiero economico, la vera questione cruciale dei tempi moderni, che accomuna pressoché tutti i Paesi sviluppati. Da ciò dipendono, in buona misura, sia le aspettative dei mercati finanziari, che conseguentemente la sostenibilità dei debiti pubblici nazionali e quindi anche le prospettive di crescita dell'economia nel quadro della congiuntura e degli equilibri dell'economia internazionale. È passato il tempo in cui valeva sempre l'equazione manovra di contenimento uguale manovra recessiva. Voglio solo sottolineare a questo punto che l'insieme delle manovre della primavera-estate comprende un decreto per lo sviluppo economico che è bene mettere subito in esecuzione. Molti non ricordano che lì vi sono delle norme che vanno implementate con rapidità. In tal senso, se per un verso appaiono indubbi e riconoscibili sin d'ora gli effetti di retroazione che la correzione può produrre, almeno nel breve periodo, va riconosciuto altresì che solo tramite questi inasprimenti e questi sacrifici, e liberandolo le energie creatrici di cui il Paese è ricco, l'Italia potrà riavviarsi su un sentiero di crescita più elevata, stabile e soprattutto duratura. È chiaro in tal senso che sin d'ora, anche al di là delle correzioni sugli andamenti tendenziali della spesa pubblica, come nel dibattito circa la iscrizione o meno in Costituzione del principio del pareggio, si imponga come prioritaria e indifferibile una riflessione sulle grandi scelte che attengono alla riduzione della presenza del settore pubblico nell'economia e alle riforme strutturali che in questo provvedimento, in tema di lavoro e di liberalizzazioni, così come in materia di *spending review* e razionalizzazione, sono comunque presenti. Occorre farlo nella consapevolezza che la quota così elevata di PIL oggi intermediata da parte del settore pubblico, attestata su livelli pari ad oltre il 50 per cento, finisce inevitabilmente per irrigidire, se non per paralizzare, il dinamismo e la crescita dell'economia nazionale. Questo stato di cose non è più sostenibile, e già il ripristino del pareggio di bilancio con un anno di anticipo che si otterrà con la correzione in esame, rispetto a quanto inizialmente stabilito con la manovra di luglio, dovrà influire favorevolmente sull'innalzamento del del tasso di crescita dell'economia, almeno a partire dal 2013. Ma, più in generale, si tratta, per quanto nella responsabilità degli indirizzi di politica economica di cui occorre oggi discutere, di valutare l'opportunità di procedere con la massima speditezza verso una più complessa ridefinizione e riqualificazione della presenza dello Stato nell'economia. Occorre, lo ribadisco, procedere verso una riduzione della sua presenza, ma anche favorire un rinnovata qualificazione del suo contenuto mediante misure di contenimento non più lineari ma selettive, tramite il potenziamento dell'azione in tutta quella gamma di infrastrutture e servizi il cui potenziamento si rende necessario per il sostegno alla crescita dell'economia. Spendere meno, dunque, ma anche spendere meglio, redistribuire il carico fiscale dal lavoro alle rendite, liberalizzare i mercati: sono gli assi portanti di questa manovra. Occorre che lo siano anche nel prosieguo della nostra azione. Naturalmente, signor Presidente, mi riservo, in seguito alla presentazione di nuove misure nell'emendamento del Governo, di integrare la relazione su quel punto. Vi ringrazio.

malgrado le novità si annuncino cospicue e rilevanti, continuo a credere (e forse ormai sarebbe meglio che dicessi che

So che ormai devo concludere che mi sbaglio, ma questo è il mio mestiere e questo cerco di fare. BALDASSARRI *(Per il

Presidente, viviamo ore drammatiche. Nessuno, nemmeno la cancelliera Merkel, può permettersi di accostare la situazione italiana a quella greca *(Applausi dal può permettersi di sottovalutare il rischio che incombe sul nostro Paese. Sì, il debito pubblico italiano può fallire, e l'insolvenza di un grande Paese come l'Italia può trascinare con sé nella rovina l'intero sistema dell'euro. Tornerò più avanti su questo punto per motivare meglio giudizi tanto allarmanti. Ora voglio concentrarmi sulle cose da fare nelle prossime ore, non sulle analisi di ciò che è stato. Il Presidente della Repubblica ieri, al termine di una giornata drammatica per il nostro Paese, ha chiesto di rafforzare l'efficacia e la credibilità della manovra. Adesso noi tutti, maggioranza, Governo e opposizione, ciascuno secondo la sua responsabilità, dobbiamo rispondere a quell'appello. Lo deve fare il Governo che ai primi di agosto aveva dato segni di una consapevolezza e di una determinazione che si sono poi, via via, affievolite, fino a tradursi in una vera e propria confusione e irresponsabile improvvisazione. I segni di consapevolezza, li voglio enumerare: la decisione di rafforzare, rispetto alla sua prima versione, la manovra di luglio; la convocazione l'11 agosto delle Commissioni bilancio e affari costituzionali per mettere all'ordine del giorno l'introduzione in Costituzione della regola sul pareggio strutturale di bilancio; il varo della manovra il 13 agosto. Ma poi, in rapida sequenza, i segni di confusione, di sottovalutazione del rischio, di incompetenza, di irresponsabilità hanno avuto la prevalenza. Confusione e sottovalutazione: se si è davvero convinti che il debito pubblico italiano può fallire, e purtroppo può fallire, inserisce nella manovra il contributo di solidarietà - per discutibile che esso sia - per poi toglierlo dopo qualche giorno, sostituendolo con i proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Cosa può capire il cittadino se un giorno il suo Governo gli dice che la casa brucia e che bisogna ricorrere ad un estintore assolutamente inusuale, capace anche di provocare effetti indesiderati molto sgraditi, e il giorno dopo quello stesso Governo gli comunica che si può fare a meno di quello stesso istituto? Il cittadino capisce che l'incendio non doveva essere poi così grave se il Governo si comporta così, e tende a comportarsi di conseguenza. Ma se il cittadino si comporta di conseguenza noi non riusciamo ad affrontare la crisi e a fare a meno di cadere nel baratro che sta di fronte a noi. L'incompetenza: prima l'annuncio di una misura in materia previdenziale che discrimina pesantemente centinaia di migliaia di lavoratori laureati che hanno onerosamente - almeno quelli che lo hanno fatto negli anni più recenti riscattato a fini previdenziali gli anni dell'università. «Poche migliaia di persone» - ecco l'incompetenza - si sente dichiarare da Ministri ai margini dell'infausto vertice di Arcore. Poi la precipitosa corsa all'indietro e ad una chiusura verso qualsiasi intervento in materia previdenziale che, a sua volta, è uno dei principali fattori di scarsa credibilità della manovra. Per non citare, signor Presidente, il danno arrecato al Paese dallo sconcertante intervento, a Cernobbio, del Ministro degli affari esteri in materia di autonome scelte della Banca centrale europea in tema di interventi non convenzionali dell'istituto di emissione sul mercato dei titoli del debito pubblico. del debito pubblico. Un intervento che ha provocato una reazione ufficiale della Banca centrale europea nel momento in cui è massimamente impegnata a fornire al debito pubblico italiano il sostegno compatibile con il suo statuto: un comunicato ufficiale per respingere sdegnosamente le sollecitazioni indebite del Ministro degli esteri del Governo italiano. Irresponsabilità, signor Presidente: se era opportuno - e forse lo era - offrire una copertura di legge all'accordo sulla rappresentanza e la contrattazione concluso il 28 giugno tra tutte le parti sociali, anche al fine di consentire ad una ben regolata e diffusa contrattazione di secondo livello di derogare al contratto nazionale (ricordiamoci che la Germania deve una parte importante del suo rilancio ad una scelta di questo tipo), qual è la ragione che ha mosso il Governo a scrivere l'articolo 8 della manovra, che produce scontro sociale e conflitto anche tra i protagonisti, anzi proprio tra i protagonisti, dell'accordo del 28 giugno?

Come è potuto accadere che, a distanza di tre settimane, il Governo non abbia depositato una precisa proposta di riforma e che le Commissioni competenti della Camera non si siano più riunite da allora fino ad oggi? Qualcuno dice non è roba che si conta, che influisce sui saldi - quella dell'articolo 81 - e ci sarà dunque tempo per provvedere. Chi sostiene questa tesi non ha ben compreso la qualità della crisi nella quale siamo immersi, signor Presidente. Questa è prima di tutto una crisi di fiducia che, deprimendo le aspettative, gela consumi e investimenti, diffonde incertezza e per questa via - come mostra da tempo l'andamento dei CDS - alimenta la previsione della possibile insolvenza.

sulla regola del pareggio strutturale di bilancio in Costituzione è merce che vale quanto e più dell'oro, nella crisi attuale. Altro che non influire sui saldi! Influisce sul merito di credito del Paese, e dunque sui tassi di interesse, più di qualsiasi altra misura. Lo dimostra la Spagna

Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, un buon livello di coesione sociale nel sostegno alle misure anticrisi è essenziale per il loro successo. Per convincersene basta guardare quanto accade rispettivamente in Grecia e in Spagna.

Dall'altra parte, in Spagna voto al 90 per cento delle Cortes sul pareggio in Costituzione e conflitto sociale più moderato. Il Paese sembra recuperare, malgrado abbia - lo sappiamo tutti fondamentali dell'economia assai più deboli di quanto non siano quelli dell'economia italiana. Questo confronto, signor Presidente, fornisce al Governo una indicazione che, giunti a questo punto, non può essere disattesa, se il Governo è responsabile. Cancelli il secondo comma dell'articolo 8 per creare quel clima di rispetto e di reciproco riconoscimento di ruolo tra le parti sociali e il Governo del Paese che è la premessa indispensabile di un buon quadro di coesione sociale. Un Governo che chiede responsabilità a tutti, che deve potersi giovare di uno sforzo collettivo, può e deve mostrare responsabilità. Sull'articolo 8 il Governo non mostra questa responsabilità; lo faccia adesso e noi gliene daremo volentieri atto. Il rischio è elevatissimo. Ma c'è ancora modo e tempo per farvi fronte, purché - ha detto il presidente Napolitano, che ancora voglio ringraziare in questa occasione - «sforzi rivolti a questo fine non vengono bloccati da incomprensioni e da pregiudiziali insostenibili». Il Paese ha le risorse per farcela. Ha le risorse di sapere, di saper fare, di voglia di fare. Ha le risorse economiche, nella potenza del suo apparato produttivo manifatturiero e nella capacità di risparmio delle sue famiglie. È ora la politica che deve mostrare di possedere le risorse necessarie per guidare il Paese, con mano ferma, verso la stabilità e la ripresa. Dal lato del Governo, per ora, è emerso un grave *deficit* di forza, di coesione, di visione, di *leadership*. Avrebbe dovuto prenderne atto e favorire la formazione di un nuovo Governo, sostenuto da tutte le principali forze politiche, di qui fino al 2013. Sarebbe così stato rimosso quello che è oggi il principale fattore della crisi di fiducia che investe il Paese: la scarsa o nulla credibilità dell'Esecutivo. contando sull'abborracciato consenso di cui tuttora gode in Parlamento, il Governo ha deciso - per usare l'espressione canonica - di andare avanti. Questa però non può rimanere, signor Presidente, l'unica decisione di cui questo Governo è capace. Andate avanti, signori del Governo? Allora, rafforzate subito la manovra, sia dal lato della stabilità, sia dal lato della ripresa economica. E fatelo adesso, perché se tra 15 giorni dovrete fare un altro intervento, allora l'Italia sarà avviata in una sindrome greca: provvedimenti, anche corretti, ad uno ad uno, e necessari, ad uno ad uno, si rivelano sempre insufficienti, perché assunti in ritardo sistematico di almeno un mese rispetto a quando sarebbero stati davvero utili e risolutivi. Dunque, la manovra va rafforzata adesso, non tra 15 giorni, perché allora sarà troppo tardi. Come rafforzarla? È difficile, signor Presidente, dall'opposizione, fare tutte le parti in commedia. È impossibile, checché se ne sia detto in passato, in particolare nel partito di cui ho fatto parte, "governare dall'opposizione": ce l'eravamo inventato perché al Governo davvero non ci potevamo non ci potevamo andare, ma governare dall'opposizione nelle democrazie normali e competitive non si può. Possiamo però, come opposizione, sollecitare e favorire una svolta, da parte di chi pretende di conservare la direzione politica del Paese. Noi, al posto vostro, signori del Governo, avremmo impostato sin dall'inizio un'altra manovra: più risparmi da revisione integrale della spesa e piano industriale della pubblica amministrazione, minore aumento della pressione fiscale. Più coraggio sulle liberalizzazioni dei mercati chiusi, a partire dal settore strategico dell'energia. Un robusto spostamento di prelievo dal lavoro - specie quello femminile e giovanile - alla rendita e ai consumi. Una violenta cura dimagrante per la politica e i suoi costi, col primo voto, già a settembre, per le riforme costituzionali necessarie a dimezzare il numero dei parlamentari e a ridisegnare l'assetto delle autonomie locali, in chiave di semplificazione e snellimento. Un intervento non di riforma della previdenza - perché quella l'abbiamo fatta nel 1995-1996 - ma di accelerazione della sua universale applicazione - col metodo del calcolo contributivo *pro rata temporis* anche tenendo conto dell'ulteriore progresso dell'attesa di vita tra il 1995 ed oggi. Un'aggressione al nodo del debito pubblico, per tagliarlo una buona volta, sia attraverso la valorizzazione e l'alienazione di quote rilevanti del patrimonio pubblico - rigorosamente destinando ogni euro a riduzione del volume globale del debito - sia ricorrendo ad una imposta patrimoniale ad aliquota moderata

posseduta dal 10 per cento delle famiglie più dotate di ricchezza patrimoniale. Una decisa lotta all'evasione fiscale, fondata sulla drastica riduzione dell'uso del contante e sul conflitto di interessi tra contribuenti,

che aggredisce contemporaneamente tutti e tre i fattori di difficoltà del Paese: eccesso di disuguaglianza, scarsa crescita, eccesso di debito pubblico.

così ciascuna di queste scelte che ho illustrato integra e rende produttiva l'altra, in modo tale che nessuna è davvero efficace fuori dal disegno organico di cambiamento che tutte le collega e le tiene assieme. Se ci aveste dato retta, già a luglio, oggi non saremmo qui a discutere sull'esigenza di rafforzare la manovra per renderla più credibile.

constatare che l'approdo raggiunto - il testo del decreto così come emendato dalla 5a Commissione - non è il posto nel quale dobbiamo arrivare per recuperare credibilità e ispirare fiducia. Noi, dato il contesto creato dalla vostra manovra, profondamente diverso da quello che abbiamo proposto, vi abbiamo tuttavia fornito, con i nostri emendamenti,

spiccano quelle per la revisione integrale della spesa pubblica e per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie - che ora aprono il testo del decreto - e sono il frutto di due proposte del Gruppo del Partito Democratico. Se il Governo Se il Governo sarà pari alla sfida contenuta in queste due norme - la legge delega sulle circoscrizioni giudiziarie e la legge sulla *spending review* - il Paese potrà trarne un enorme giovamento, sia per l'accresciuta efficienza economica, sia per la riduzione e la qualificazione della spesa. Ma queste due rilevantissime riforme strutturali non hanno il potere di trasformare questa manovra in altro da sé. Essa resta troppo debole (troppa parte delle maggiori entrate è incerta) e squilibrata (nessun intervento per la crescita, eccessivo aumento della pressione fiscale). È vostro preciso dovere rafforzarla con misure strutturali di riduzione, nel medio-lungo periodo, della spesa e di riequilibrio della pressione fiscale tra lavoro e impresa, da una parte, e altre basi imponibili, dall'altra. È quello che vi chiediamo dall'inizio. È quello che dovete dovete fare. Misure che noi vi chiediamo di assumere, ma di cui voi vi dovete assumere pienamente la responsabilità politica. Il nostro giudizio, su ognuna di esse, quando le vedremo, sarà direttamente proporzionale alla distanza che separerà che separerà ciascuna scelta rispetto alla strategia alternativa che noi vi abbiamo proposto e che voi avete rifiutato. Su ognuna delle scelte siamo pronti ad un confronto di merito, punto per punto, come abbiamo fatto durante il lavoro della 5a Commissione, senza avanzare pregiudiziali, come ci ha chiesto il Presidente, e sempre ribadendo l'alternatività del nostro disegno di fuoriuscita dalla crisi. Quanto al resto, dovete depositare subito alla Camera un disegno di legge di riforma costituzionale sull'articolo 81, cosicché si possa discutere e decidere in pochi giorni, prima alla Camera e poi al Senato. E decidetevi una buona volta: se avete una vostra proposta sull'articolo 81, presentatela entro domani. Se non l'avete, consentite che si proceda all'esame dei disegni di legge già presentati. Dovete, infine, consentire che Camera e Senato votino subito per dimezzare il numero dei parlamentari. Se non siete in grado di fare nulla di tutto ciò - e restate bloccati dai veti di questa o di quella componente della maggioranza - allora prendetene subito atto, per il bene del Paese. Un nuovo Governo ad amplissima base parlamentare, cui non faremo certo mancare il nostro convinto appoggio, potrà a quel punto formarsi e guidare il Paese nel tempo che ci separa dalle elezioni del 2013. Chiedo infine, signor Presidente,

signori del Governo, colleghi, è una sorta di commedia degli equivoci quella che si sta sviluppando nell'Aula del Senato, perché non sappiamo su quale testo stiamo avviando la discussione. Non sappiamo se è quello uscito dalla Commissione bilancio oppure se è quello che è stato annunciato a mezzo stampa, tramite le agenzie. Non sappiamo se verrà aumentata l'IVA, la tassa sui poveri, né se ci sarà una patrimoniale. Insomma, signor Presidente, ci auguriamo che questa manovra

i depositi delle banche alla BCE sono volati a 166,8 miliardi di euro, uno dei massimi storici;

Ciò, signor Presidente, perché vi è una crisi profonda: non solo quella sistemica dei mercati, infarcita di finanza di carta che alimenta la speculazione, colpisce le imprese, i lavoratori e le famiglie, attacca la sovranità degli Stati e detta la propria agenda alla politica, ma quella irreversibile di un Governo e di una maggioranza commissariati dalla Banca centrale europea; un Governo che annaspa nel buio e non offre alcuna soluzione credibile ai problemi di un grande Paese come l'Italia. Siamo stati facili profeti, signor Presidente, quando nel corso della discussione dell'ultima manovra, approvata circa un mese fa, avevamo avvertito che occorrevano misure più decise e strutturali ed una stagione di riforme per aiutare le famiglie, le imprese ed i cittadini ad uscire dalla crisi. Ma l'autosufficienza di Governo e maggioranza non ha voluto neppure prendere in considerazione alcune delle proposte da noi avanzate. Anche in questa manovra, imposta dalla BCE, abbiamo avanzato proposte emendative, che avete bocciato, per migliorare testi e contenuti di un provvedimento che va a colpire i soliti noti. Noi oggi eravamo in piazza con chi rivendicava i propri diritti, intaccati da questo articolo 8: lo Statuto dei diritti dei lavoratori che è costato lacrime e sangue a intere generazioni. Noi eravamo in piazza e rivendichiamo i diritti della gente a protestare contro una manovra che non colpisce gli gli evasori, i riciclatori di denaro sporco e i faccendieri che hanno prosperato negli ultimi tre anni. Uno Stato di diritto, come non fa accordi con la mafia e la criminalità organizzata, non può scendere a patti con riciclatori di denaro sporco ed evasori che sottraggono dai 120 ai 130 miliardi di euro all'anno dall'imponibile. Ciononostante, sono stati condonati dal ministro Tremonti con un'aliquota del 2,5 per cento nel 2003 e del 5 per cento nel 2009 per il rimpatrio virtuale di capitali esportati illecitamente all'estero, lavati in forma anonima nella grande lavanderia statale con un vero e proprio riciclaggio di Stato e riportati in gran parte nei paradisi fiscali. Avevamo proposto un'imposta patrimoniale del 20 per cento su 105 miliardi di euro scudati che, oltre a far pagare per la prima volta evasori e riciclatori, avrebbe fatto rientrare nelle casse dello Stato 21 miliardi di euro per compensare il taglio dei trasferimenti agli enti locali, impedendo attacchi a pensioni e Stato sociale, consentendo di eliminare i *ticket* sulla salute e l'aumento delle accise sui carburanti, impedendo che i risparmiatori che sono stati truffati dalle banche (con le quali il Governo continua ad andare a braccetto) oltre al danno debbano subire la beffa di pagare i bolli su custodie di titoli andati in fallimento. Non esistevano ostacoli, né tecnici né giuridici, e non esisteva la violazione del sacro principio dell'anonimato. Voglio ricordare che altri Paesi più seri, quando fanno gli accordi

che sono stati evasi ed elusi, le banche gli intermediari che avevano riportato quei capitali possono fare da sostituti d'imposta e non si sarebbe violato il principio sacro dell'anonimato, ammesso che quelli che hanno vissuto come tenie nel corpo dei contribuenti onesti debbano anche avere garantito l'anonimato. Avevamo proposto che alcuni boiardi di Stato, che prendono doppi stipendi di 400-500.000 euro l'anno, oltre ai *benefit*, potessero rinunciare ad uno uno di essi. Milena Gabanelli in una puntata di «Report» aveva individuato questi signori che prendono doppi stipendi. Avevamo proposto di eliminare gli scandalosi collaudi ed arbitrati dei giudici amministrativi,

Avevamo proposto l'abolizione dell'odiosa commissione di massimo scoperto (una vera e propria taglia sugli impieghi per retribuire gli stipendi dei banchieri), una patrimoniale sui patrimoni, il divieto di domiciliare imprese a partecipazione pubblica nei paradisi fiscali e/o legali per eseguire operazioni non sempre pulite, un contributo straordinario sui calciatori, l'inasprimento della tassazione sulle bevande gassate, che procurano seri danni alla salute, come ha fatto il presidente francese Sarkozy. sul conflitto di interesse tra prestatore d'opera e utente che, potendo detrarre dalla dichiarazione dei redditi una parte fino a 2.000 euro delle prestazioni ricevute, avrebbe fatto emergere l'evasione fiscale. Avevamo proposto una tassazione sui fissati bollati per arginare *trading* speculativi, nonché contenitori più conformi alle confezioni dei farmaci per evitare sperperi e sprechi di medicinali, che ricadono sulla spesa 18,30)** (*Segue* LANNUTTI). Signora Presidente, in una fase di turbolenza dei mercati e della speculazione sistemica avevamo proposto il divieto delle vendite allo scoperto per impedire che si possa speculare in borsa scommettendo sui ribassi senza neppure avere il possesso dei titoli. Avevamo proposto il divieto di emettere *report* sull'Italia da parte delle cosiddette tre sorelle del *rating* - Moody's, Standard & Poor's e Fitch - fino a quando non ottengano la registrazione da parte dell'ESMA, l'autorità di borsa comunitaria che ha bocciato le richieste di queste agenzie. Avevamo proposto la vendita dell'oro di Bankitalia (che - voglio ricordare - non è del signor Draghi, né di *monsieur* Trichet,

è arrivato a 1.901,9 miliardi, crescendo più con i Governi di centrodestra che con quelli di centrosinistra. Negli ultimi mesi esso è aumentato di 6,4 miliardi al mese, rispetto ai 3,9 miliardi dei precedenti Governi. Altro che eredità del passato! Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. È arrivato il momento che gli Stati democratici riuniti nel G20, sotto scacco dei mercati di carta, di banche di affari, fondi speculativi, banchieri, oligarchi e leve finanziarie fondate sull'azzardo, che hanno contagiato l'economia reale fatta di sudore e lavoro, ritrovino la giusta rotta, rifiutando la dittatura di speculatori professionisti agenzie di *rating* che hanno provocato la crisi sistemica e corroso la sovranità degli Stati, prosciugando i risparmi e distruggendo 32 milioni di posti di lavoro solo negli ultimi anni. Concludo affermando,

ricattano gli Stati e attentano alla sicurezza delle Nazioni e alla sovranità degli Stati. Non c'è nulla di tutto ciò da parte di questo Governo e, per questa ragione, rivendichiamo di essere stati in mezzo ai lavoratori che hanno scioperato oggi, perché difendiamo i diritti della povera gente, a differenza vostra,

Signora Presidente, colleghi senatori, da quanto offre lo scenario del confronto politico sulla manovra, Governo e opposizione ci appaiono dotati di prodigiose qualità: l'uno riuscendo fino a questo momento a preservare il Paese dagli effetti maggiormente deleteri di una crisi che travaglia l'intero vecchio continente e, l'altra, ottenendo finalmente di far spirare anche al di qua delle Alpi il vento furioso di indignazioni ben più comprensibili altrove. La propaganda incendiaria da spargere su un fuoco che da noi sembrava lungi dall'attecchire sfrutta cinicamente la paura più diffusa quando il futuro appare meno roseo e il presente si mostra denso di incognite. Parlo del timore di perdere la sicurezza economica garantita dal posto fisso di lavoro: apprensione che certa parte politica alimenta esacerbando gli animi. Il livello di questa operazione strumentale si esprime pienamente nella parola d'ordine lanciata da un esponente di primo piano dell'opposizione. Cito testualmente: «Il Governo odia gli operai». una sentenza proveniente dalla parte politica che ha spalancato e vorrebbe ancor più spalancare le porte all'immigrazione per offrire il regalo più gradito al grande capitale:

Quale credibilità può essere attribuita a simili paladini dei lavoratori, quando si stracciano le vesti per le presunte iatture conseguenti alle modifiche all'articolo 8 della manovra? Dove mai ravvisano costoro l'automatismo tra il trasferimento della contrattualità a livello aziendale o territoriale e le agevolazioni al licenziamento? Forse non risulterà sufficientemente esplicito il testo di questa misura pensata per imprimere maggior dinamismo al sistema produttivo, e dunque per favorire la crescita; evidentemente esso si presta a speculazioni e a strumentalizzazioni, ragion per cui necessiterebbe di una migliore esposizione. Eppure, nella sua interpretazione mi parrebbe serio attenermi alla linea guida fornita dal ministro del lavoro Sacconi, il quale chiarisce che per il provvedimento in discussione «non ha senso parlare di libertà di licenziare o usare altre semplificazioni che non corrispondono, neppure lontanamente, alla oggettività della norma». Giova al riguardo anche la delucidazione di Michele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro presso l'università degli studi di Modena. Il giuslavorista garantisce - cito testualmente - che «il decreto non dà nessuna libertà di licenziamento», e che «gli accordi non possono derogare al divieto di licenziamento senza giustificazione. Possono semmai, in casi specifici, prevedere norme diverse rispetto al reintegro, che peraltro c'è solo in Italia». D'altro D'altro canto, mi chiedo su quale pianeta vivano quanti strillano di Statuto dei lavoratori calpestato e di Costituzione violata per la presunta facoltà di licenziare introdotta dalla manovra. Ci rendiamo conto di quante siano le aziende che si sbarazzano di intere unità produttive e delle relative maestranze e delocalizzano all'estero, quasi fosse la cosa più naturale del mondo? Perché chi adesso strilla contro la presunta libertà di licenziamento non si è mai scagliato con tanta veemenza contro quegli imprenditori, magari illuminati e progressisti, che tolgono il lavoro ai nostri operai per darlo ai cinesi? È precisamente in questi casi, purtroppo sempre più frequenti, che la contrattazione locale ed aziendale già oggi interviene a mitigare le conseguenze della perdita del posto, e a nessuno appare come una minaccia ma piuttosto come una scialuppa di salvataggio, una risorsa. Confidiamo pertanto che questo aspetto della manovra giunga ad istituzionalizzare tali meccanismi, a maggiore tutela dei lavoratori. La verità è che, a dispetto degli *spot* di qualcuno sulla virtuale questione della libertà di licenziare, la posta concreta e di maggior rilievo dell'attuale manovra era ed è un'altra. Si tratta delle pensioni, si chiama Lega Nord la forza politica che non è arretrata di un passo rispetto alle sue posizioni, salvaguardando ancora una volta i diritti maturati dai lavoratori. Per non toccare le pensioni, a suo tempo la Lega lasciò un Governo e una maggioranza: a questa determinazione non rinunciamo neppure ora che alcuni interpretano nel senso di un intervento sul sistema pensionistico l'esortazione del Capo dello Stato ad attuare provvedimenti di maggiore impatto. Da parte nostra, fatichiamo a cogliere l'urgenza di un ulteriore inasprimento della manovra-*bis*, che già prevede interventi per circa 45 miliardi e che, sommata alla precedente da 47 miliardi, varata dal Governo a fine giugno, supera la quota *record* dei 90 miliardi di euro. decreto all'esame possegga i numeri per centrare l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, sollecitato dalla BCE, senza bisogno di allungare le mani sulle pensioni. A garanzia A garanzia dell'efficacia della manovra restano i capisaldi di un sempre più fruttuoso recupero dell'evasione fiscale, a cui si aggiunge la prospettiva concreta del carcere per i grandi evasori e dei tagli che indurranno ad una maggior oculatezza gli amministratori degli enti locali, i quali lamentano il calo delle risorse per i servizi di carattere sociale ma, in troppi casi, non rinunciano a largheggiare in manifestazioni, feste, strapagati consulenti e spese del tutto opinabili. Nel complesso, dunque, assistiamo a interventi di portata estremamente significativa, che una volta compresi otterranno la condivisione dei cittadini con la testa sulle spalle. Interventi che specularmente provocano la pregiudiziale avversione di chi antepone il calcolo di parte all'interesse collettivo, al punto da organizzare scioperi che costano miliardi di euro al Paese.

credo che dovremmo partire proprio dall'auspicio che il presidente Schifani ha rivolto all'Aula all'inizio della seduta alla quale stiamo partecipando, quello cioè di approvare rapidamente la manovra al nostro esame, ma immagino che ogni collega in questo momento si ponga il problema di capire quale manovra stiamo approvando, tale e tanta è stata la confusione che ha caratterizzato questi giorni e queste ore che ci lasciamo alle spalle. Devo ringraziare sinceramente il Presidente della Commissione bilancio, il senatore Azzollini, e il relatore di minoranza, il senatore Morando, per lo sforzo che hanno compiuto di illustrare una manovra che probabilmente domani mattina non ci sarà più. Infatti, quale manovra saremo chiamati ad approvare? Quella del contributo di solidarietà a carico dei dipendenti pubblici o quella dell'abolizione, ai fini del computo degli anni per il godimento della pensione, del riscatto degli anni di studio universitario o del servizio militare obbligatorio, o quella della patrimoniale mille volte smentita ma domani probabilmente inserita nell'emendamento *omnibus*? O ancora quella dell'IVA, che il Ministro dell'economia osteggia, ma che anch'essa probabilmente troveremo domani quale suggello definitivo della confusione che ha caratterizzato l'iniziativa del Governo? O quella ancora della lotta all'evasione, che si arresta timidamente ai confini della Svizzera, lì dove invece altri Paesi pressano in maniera decisa per scoprire i capitali imboscati nelle banche di quel Paese? O ancora sarà la manovra che non metterà le mani nelle tasche degli italiani, come ha più volte ribadito il Presidente del Consiglio, o non sarà invece la manovra che metterà le tasche degli italiani nelle mani degli speculatori, quegli stessi speculatori che quotidianamente impoveriscono le nostre Borse e quotidianamente fanno lievitare i differenziali tra i buoni del Tesoro italiani e i *Bund* della Repubblica tedesca? Questo è il dilemma che quest'Aula ha di fronte, accanto ad un dilemma ancora più drammatico, quello dell'utilità del lavoro delle Assemblee parlamentari. non è la prima volta che capita in questa legislatura di assistere ad una scena ormai stantia, quella di una Commissione, sia essa la Commissione bilancio sia essa la Commissione giustizia, che lavorano per giorni, per ore, a volte anche di notte, per mettere a punto provvedimenti fondamentali per il rinnovamento del Paese, per il consolidamento delle sue finanze, e poi, quando il provvedimento precipita in quest'Aula, ci si trova di fronte alla solita apposizione della fiducia che il Governo ripetutamente introduce per annichilire qualunque dibattito e qualunque confronto tra le diverse posizioni presenti anche in questa circostanza.

che abbia proprio nella vastità del consenso espresso quell'autorevolezza che i mercati invocano, che i mercati attendono; un

dalle secche di un'instabilità per troppo tempo sopportata e per troppo tempo tollerata. Concludo, signora Presidente, ricordando soltanto i punti attraverso i quali un Governo degno di questo nome, consapevole della difficoltà della situazione che è chiamato ad affrontare, avrebbe dovuto definire una manovra di tale portata, attraverso provvedimenti strutturali, misure per la crescita, riforme strutturali, che cito soltanto per titoli avendo oramai consumato il tempo a mia disposizione. Una riforma della pubblica amministrazione per tranciare definitivamente i lacci e lacciuoli che si frappongono alla libera iniziativa e al vivere civile dei cittadini; una riforma fiscale in grado di rompere quel circolo vizioso fra carico fiscale ed evasione; una riforma della giustizia; una riforma istituzionale che ponga fine al bicameralismo perfetto ed elimini tutti gli orpelli istituzionali di uno Stato pesante, le Province, gli enti inutili; le liberalizzazioni e le privatizzazioni; inoltre, una questione accantonata nel dibattito non soltanto di queste ore, ma nel dibattito che ha caratterizzato la manovra, ossia la questione di un Mezzogiorno che non può essere abbandonato a se stesso, che va integrato nella nella crescita, nello sviluppo di questo Paese pur all'interno di questa nuova cornice federalista della quale tanto si parla, ma che viene negata con provvedimenti assolutamente insufficienti e parziali. Di ciò avrebbe avuto bisogno il Paese; di questa manovra avrebbero avuto bisogno gli italiani; di simili assicurazioni avrebbero avuto bisogno i mercati. Credo che domani ci troveremo di fronte all'ennesima farsa che produrrà ulteriori guasti

senatori, è con qualche imbarazzo che prendo la parola in questo dibattito su un oggetto che ancora non conosciamo, di fronte a un'Aula più vuota del solito. Penso che se fossi andato nelle aule che frequentavo fino a qualche anno fa, dopo aver precisato ai miei studenti che il giorno dopo avrei presentato il vero programma del corso e che quel giorno avrei fatto lezione su un argomento che non rientrava nel programma d'esame, probabilmente avrei ottenuto lo stesso risultato. forse cominciare dal metodo, perché c'è un po' di follia in questo metodo: così direbbe Polonio se invece che nella tragedia di Amleto si fosse trovato nella *pièce* che stiamo recitando qui oggi. Dopo la manovra di luglio, approvata in pochi giorni su sollecitazione del Capo dello Stato, questa di agosto nasce già legge con un decreto-legge del 13 agosto, e poi vive subito una serie di disconoscimenti di paternità sulle varie norme che sembrano da pochi o da nessuno condivise, da pochi o da nessuno volute. Questa manovra vive una serie di aggiornamenti non frutto di lavori parlamentari di una Commissione, che peraltro ha bene e molto lavorato nella settimana che si è appena conclusa, ma di vertici un po' improvvisati a casa di questo o di quello, dove apprendiamo di un testo 2 il giorno 29, di un testo 3 il giorno 30, svariate altre novità nella settimana in cui la Commissione lavorava, ma non emerse dall'aula dalla Commissione, bensì da fuori di essa. Poi, all'atto finale di quella che doveva essere la discussione in Aula del provvedimento infine partorito dai lavori della Commissione, ci viene detto che il provvedimento verrà presentato domani, ma per quello che valgono i lavori di quest'Aula possiamo benissimo portarci avanti con il lavoro e parlare un po' a vuoto. bene ha fatto chi ha lasciato l'Aula per protestare contro questa situazione. E in questo cambiamento di testi, di posizioni, di proposte e di controproposte, nel corso di queste due settimane abbiamo visto e sentito di tutto: la supertassa chiamata eufemisticamente «contributo di solidarietà», che è andata e venuta e che forse domani tornerà; «le pensioni sì», «le pensioni no», e poi alla fine quell'ipotesi - per fortuna poi subito abortita della truffa a chi ha riscattato gli anni dell'università e del servizio militare; «l'IVA sì», «l'IVA no», e poi la geniale e surreale battuta dell'IVA a tre mesi,

una manovra economica che fosse non soltanto efficace per il Paese, ma credibile per il mondo, ebbene, da questo punto di vista abbiamo completamente fallito, abbiamo fallito ce lo stanno dicendo in queste ore i mercati, che non sono i cattivi dei film, come qualcuno li vuol fare apparire. I mercati sono la sintesi del giudizio degli operatori internazionali sulle prospettive future della nostra economia e quindi, in larga parte, sulle capacità presenti non già della nostra economia, ma della nostra politica. Spesso infatti i mercati valutano positivamente un'economia debole, emergente, in costruzione, se è presente un chiaro progetto per il futuro, una forte volontà di realizzarlo e una classe politica che antepone il bene del Paese alla propria sopravvivenza o alla propria progressione. È esattamente il contrario di quanto avviene in Italia. Il nostro è ancora un Paese abbastanza ricco, forse siamo intorno al decimo posto

scivolati nella parte bassa della classifica per tutti quegli indicatori che influenzano il futuro economico e civile di una società, tra cui certamente il tasso di crescita, ma anche la competitività, gli investimenti diretti esteri, la trasparenza,

ed è ai primissimi posti nel mondo (terzo o quarto) per debito pubblico, o è anche ai primissimi posti come modello internazionale per la produzione e la qualità di beni e servizi pubblici (dall'assistenza alla scuola, dalla sanità alla giustizia, dalla ricerca alle infrastrutture), oppure, se non è così,

che poi non ha mai attuato. Ecco quindi le considerazioni sul merito. Anche questa manovra, come quella di luglio, insegue con sempre maggiori entrate quella che è in realtà la sempre maggiore spesa, che è il vero costo della politica, e definisce tagli quelli che invece sono rallentamenti nella crescita della spesa: esattamente il contrario dello spirito liberale che l'attuale maggioranza si proponeva di portare nel Paese. E da dove mai sarebbe dovuta una rivoluzione liberale dell'Italia, se non da una seria ed equa riforma della fiscalità, con un fisco finalmente giusto e anche severo, che recuperasse almeno in parte quei 130 miliardi di gettito evaso

quando il Paese è in crescita, queste si tollerano, dal momento che ognuno è intento a contemplare il proprio benessere, ma quando il Paese è in recessione, diventano insopportabili, perché ognuno guarda al benessere altrui. vera riforma del fisco, dunque, avrebbe dovuto rendere i cittadini, se non felici di pagare le tasse, almeno convinti e consapevoli che ciò serve al benessere del Paese e delle future generazioni e non a continuare ad ingrassare le molte caste che in questo Paese esistono, non fornendo alibi per non pagare le tasse, come si Pertanto, anche quella sovrattassa, quel contributo di solidarietà, sparito ma che poi forse ricomparirà, non avrebbe toccato loro, come loro, come non avrebbe toccato i grandi patrimoni, così come non avrebbe toccato le rendite finanziarie, portate sì al 20 per cento, ma che in nessun modo possono contribuire a raggiungere quella soglia

Einaudi diceva che l'imposta patrimoniale è iniqua, partendo dal presupposto che il patrimonio fosse frutto di una costituzione legittima in cui si sono pagate le imposte sui redditi; oppure, che fosse stato ereditato attraverso il filtro di una generosa imposta di successione. Ma nel Paese dove l'imposta di successione non esiste e le imposte sui redditi sono così spesso evase, il patrimonio spesso è frutto di una sua illegale costituzione e, spesso, questa è addirittura sancita da uno dei tanti condoni e scudi con i quali lo Stato cancella il reato, a condizione di ricevere una piccola parte della refurtiva, come faceva, in un delizioso racconto di Camilleri di qualche anno fa, un vescovo (di molti secoli fa, naturalmente) nei confronti di chi commetteva un furto, e che però poi andava a confessarsi. Si è preferito, invece, presumere che le imprese che conseguono perdite negli ultimi difficili anni siano, per definizione, delle società di comodo in mano ad evasori, lasciando loro la difficoltà e i costi e i disagi di dimostrare il contrario; si è preferito inasprire, anche in modo abnorme, le pene per gli evasori, ben sapendo che quello che conterebbe sarebbe la certezza della pena, mentre qui, invece, vi è piuttosto la quasi certezza dell'impunità. Quanto alla spesa pubblica, questo Paese è da molti anni in avanzo primario. Ciò significa che, in realtà, il *deficit* è minore del costo per gli interessi passivi sul debito accumulato negli anni precedenti. Allora è su quel debito che bisognava incidere attraverso, finalmente, un serio programma di vendita del patrimonio pubblico nelle sue varie componenti, ed è sul quel tasso di interesse che bisognava cercare di incidere per ottenere lo stesso risultato. In questo senso, si è persa l'occasione, consentitemi l'espressione un po' cinica, di questa crisi, per ottenere una vera riforma, anche sul lato della scuola pubblica. Concludo, signora Presidente, per dire che, al di là delle variazioni che saranno apportate domani mattina, e che ancora non conosciamo, nel suo impianto attuale questa manovra appare assolutamente insoddisfacente rispetto agli scopi che si prefigge.

Signora Presidente, io ho sentito sollevare diverse critiche, anche all'inizio di questo dibattito, sul metodo e sull'azione che il Governo ha posto in atto, e sta ponendo in atto, per far fronte a quella che è una difficoltà finanziaria globale, che parte da lontano, forse anche da una rivisitazione che dovremmo fare sui modelli di sviluppo, di qualità della vita e anche di Stato sociale, che dovranno essere messi in atto

stanno raggiungendo livelli di sviluppo e anche di ricchezza sempre crescenti. Abbiamo visto che si sta sviluppando, di fronte al blocco del famoso G8, anche un interessante gruppo dei Paesi BRIC, che stanno creando una contrapposizione e una alternanza anche per quelle che sono le politiche di natura economica e internazionale,

soluzioni anche diversificate, che magari in parte possono sembrare contrapposte per affrontare una situazione molto complessa e complicata al livello non solo nazionale, ma anche internazionale. Questo - a mio avviso - sta anche a testimoniare un'apertura, una capacità dialettica ampia,

dobbiamo anche rispettare i processi della democrazia. Questo Governo è stato legittimamente eletto. Questa maggioranza è ampia nel Paese

Abbiamo assolutamente la consapevolezza e la volontà di arrivare al vincolo del pareggio di bilancio, e sono assolutamente d'accordo che debba essere inserito anche in Costituzione. Mi pare stia partendo

Signora Presidente, colleghe e colleghi, prima del decreto-legge n. 98 del luglio scorso, l'indebitamento netto tendenziale

Praticamente questo significava che il nostro Paese aveva un tenore di vita più alto quasi del 4 per cento rispetto a ciò che avrebbe potuto permettersi.

Nella manovra che stiamo discutendo il pareggio si anticipa al 2013. Tuttavia, con la manovra di luglio l'Italia aveva comunque definito un percorso per mettere i conti a posto, con una clausola di salvaguardia peraltro molto forte, che prevedeva e prevede - rimanendo clausola di salvaguardia, per il sistema italiano un intervento sulle agevolazioni fiscali, qualora non fosse intervenuta la riforma del sistema delle agevolazioni e dell'assistenza, con un automatismo di taglio lineare che, fatto puramente matematico, è di oltre 32 miliardi; si tratta, quindi, di una cifra notevole. Cosa è successo? Tanti se lo chiedono. Siamo in una realtà dove la Grecia è praticamente al *default*, con tassi di interesse che viaggiano tra il 20 e il 30

il fatto che 350 milioni di europei, più qualche centinaio di migliaia di analisti mondiali, non si erano accorti che i bilanci di quel Paese non erano a posto (sono in Parlamento e, parlando di un altro

L'Europa non cresce e anche quella che fino a un mese fa era chiamata la locomotiva tedesca si è fermata; in Germania l'economia si ferma, si ferma, il cancelliere Merkel è in difficoltà e perde le elezioni e le banche tedesche sono le maggiori creditrici su Grecia ed Irlanda, che ha il grosso delle scadenze a settembre-ottobre. Un commentatore, in un articolo di fondo, questa mattina diceva che «l'irrazionalità dei mercati finanziari è evidente. Nelle quotazioni dei titoli di Stato di ieri a prestare soldi alla Germania ci si perde - un rendimento sotto il 2 per cento non copre l'inflazione - mentre a prestare all'Italia ci si guadagna più del 5,5 Il paradosso nasce dal timore che solo dalla Germania i capitali tornino indietro interi; mentre una rottura dell'euro renderebbe impossibile all'Italia pagare i propri creditori. La medesima ipotesi di catastrofe produce altri numeri ripugnanti al buon senso: sul mercato dei famigerati *credit default swap*, l'insolvenza dello Stato francese viene reputata meno remota di quella del Perù. La speculazione, naturalmente, fa affari d'oro. Il rifugio sono l'oro e i titoli tedeschi. C'è chi paventa una spaccatura dell'area dell'euro chi parla di "euromarco". Non credo, e non spero, perché - permettetemi di manifestare tutti i dubbi - se il debitore fallisce, chi paga il prezzo più alto è il creditore. L'Europa è la grande assente. Mai come ora si è manifestata l'assenza di una *governance* politica europea che valuti nell'interesse complessivo e non su dati di egoismo nazionale,

per la riorganizzazione, l'efficienza del servizio ai cittadini e la diminuzione dei responsabili di servizio, che invece l'integrazione di stipendio la portano a casa. C'è poi un intervento sulle pensioni, che probabilmente vedrà un rafforzamento, accelerare la normalizzazione del sistema pensionistico. Poi le misure sulle festività e sul lavoro. sull'esame del Documento di economia e finanza dell'Unione, che ponevano il problema della flessibilità del lavoro o del sistema dualistico italiano come uno degli elementi fondamentali.

Il Governo e la maggioranza lo hanno fatto, aperti a discutere e a confrontarsi in ogni sua parte. Il dibattito che ne è scaturito è stato vivace in maggioranza e nell'opposizione.

proposte di merito, come raccomandato dal presidente del Senato Schifani, e non solo quindi di parte, con valutazioni di maggioranza o di opposizione, che hanno avuto una valenza politica, quantitativa e qualitativa.

e non un codice di riforma, così come la clausola di salvaguardia del vecchio decreto ed anche le tante proposte che vengono in merito alla dismissione del patrimonio pubblico sono azioni tali da garantire al sistema internazionale la capacità del nostro Paese di pagare i debiti e agli italiani di salvaguardare le conquiste sociali fatte in tanti anni ed il patrimonio. Mi permetto un'ultima considerazione, come Capogruppo in Commissione bilancio del PdL, di ringraziare il presidente Azzollini, tutti i colleghi, di opposizione e di maggioranza, il presidente Schifani, venuto due volte in Commissione a

discutendo una cosa che ancora è da definire. Ovviamente intendiamo usare il nostro tempo, quello che ci è dovuto, per discutere le nostre opinioni sulla manovra, quando il Governo avrà presentato le sue innovazioni,